il tema del voto per delega dei senatori a vita nell'ambito delle Commissioni parlamentari. Tale problema si evidenzia, in queste ore e in questi giorni, con il voto quasi contemporaneo dei pareri sul Documento di programmazione economico-finanziaria e vede molto spesso determinanti i voti dei parlamentari che hanno sostituito i senatori a vita, i quali - possiamo dire - sono inconsapevoli di ciò.

una ragione in più nel caso del senatore a vita, del quale individuiamo tutti l'assoluta unicità (trattasi di un'alta personalità che, per i meriti acquisiti, è individuato dal Capo dello Stato

fosse per creare una sorta di scambio tra un'attenzione meno vigile sui conti pubblici del nostro Paese... PRESIDENTE. Vuole fare una domanda, ora dà anche la risposta? No.

sostanzialmente un emendamento molto importante perché di fatto vanifica in larga parte anche quel timidissimo tentativo di separazione delle funzioni che Commissione giustizia avevano osato introdurre nel testo, sollevando le ire dei loro maestri e mentori dell'Associazione nazionale magistrati) ha parlato di una riformulazione.

in tal caso sarebbe interessante vedere il testo e capire se è veramente una riformulazione e capire cosa pensa la Presidenza della sua ammissibilità - o se si riferiva al testo 2 già

su una notizia data dai telegiornali di oggi e che ritengo sia particolarmente seria e preoccupante: mi riferisco agli atti di vandalismo e alle minacce di tipo mafioso nei confronti dell'istituto intitolato a don Pino Puglisi, vittima della mafia, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Questi atti, che hanno comportato danni molto gravi e intimidazioni nei confronti del personale scolastico,

le attività di educazione civica e sociale antimafia che si svolgono presso l'istituto del quartiere Brancaccio di Palermo. Credo che sarebbe cosa buona

credo di aver capito la domanda del senatore Castelli, ma poiché lavoriamo sempre in questo brusìo, può anche darsi che mi sbagli e lui mi correggerà. La sua richiesta si riferisce

Quello è il testo al quale mi riferivo nel mio intervento e il collega Castelli dovrebbe averlo già ricevuto da questa mattina poiché la data che lo stampato reca è dell'11 luglio.

Voglio innanzitutto ricordare a questa onorevole Assemblea che oggi ricorre l'anniversario della morte dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, che io ho conosciuto personalmente e che, come tutti ricorderanno, fu ucciso perché era un ottimo avvocato e un ottimo servitore dello Stato. Quindi, proprio in questo momento in cui stiamo discutendo di avvocatura e di magistratura voglio dire che da parte mia e di tutti i magistrati c'è sempre stata grande considerazione e soprattutto grande apprezzamento per l'opera prestata dagli avvocati e in particolare dagli avvocati come Giorgio Ambrosoli. Per quanto riguarda

perché ne abbiamo discusso anche in sede di Comitato ristretto e di Commissione. Mi rendo conto e comprendo le ragioni che lo hanno spinto

La mia grande preoccupazione è sempre stata che questi attacchi potessero influire sull'indipendenza della magistratura, che è un bene non della categoria ma di tutti i cittadini, tant'è vero che i nostri Costituenti si preoccuparono, come prima cosa, di assicurare l'indipendenza sia alla magistratura giudicante che a quella requirente. A tale proposito, faccio presente a tutta l'Assemblea che l'indipendenza assicurata alla sola magistratura giudicante sarebbe inutile senza l'indipendenza del pubblico ministero: non credo, infatti, che, se il pubblico ministero non fosse indipendente, la magistratura giudicante avrebbe mai occasione di dimostrare la propria indipendenza.

solamente dire, proprio per la comprensione che ho essendo stato uno dei più strenui difensori dell'indipendenza della magistratura (tanto più che una magistratura indipendente risulta veramente indispensabile ad uno Stato democratico), che ho apprezzato lo sforzo che ha fatto il senatore Brutti per non far sentire alla magistratura la sensazione di una persecuzione

Se lei non lo sa, senatore Sacconi, ho rischiato anche la mia pelle per servire lo Stato, e per servirlo degnamente.

Allora, proprio per questa ragione, signor Presidente, proprio perché la magistratura pare che in questo momento abbia sentito come una persecuzione alcuni atteggiamenti - e badate che nel mio precedente intervento ho sempre apprezzato e ho fatto menzione dell'apprezzamento completo che ho avuto per i componenti avvocati della Commissione giustizia, che ringrazio ancora per il lavoro che insieme abbiamo potuto svolgere con molta tranquillità, con molta più tranquillità di quello che succede in quest'Aula

Presidente, non vorrei che si riprendesse la seduta come se si fosse sospesa con un andamento naturale. C'è stata una richiesta da parte del Ministro della giustizia di un approfondimento. Tutti sanno perfettamente che verrà presentata - anche se il presentatore non l'ha confermato - una riformulazione, a cui credo stesse dando qualche suggerimento il collega Io non ritengo si possa riprendere l'esame dell'articolo 2 quando il punto sostanziale non è ancora stato oggetto di un testo che è stato distribuito all'Aula. Senatore Calderoli, i punti sostanziali formalmente non esistono; esistono gli emendamenti che vanno discussi ordinatamente uno dopo l'altro.

Signor Presidente, intervengo su una delle tre parti su cui si è articolato l'intervento

- mi deve perdonare, Presidente, ma faccio grande fatica a rispettare l'obbligo di rivolgermi a lei e non ad altri colleghi - non mi sfugge il messaggio che l'ex autorevole esponente dell'Associazione nazionale magistrati ha rivolto alla sua maggioranza e al senatore Brutti che da qualche tempo ne pare il ventriloquo più autorevole. Mi è toccato, nel corso di questi anni, più volte intervenire a ricordo e a commemorazione dell'avvocato Ambrosoli e per questo non posso che ringraziare il senatore D'Ambrosio che oggi se ne fa promotore. Mi associo alle sue parole, ricordando la memoria di un avvocato valoroso, che è stato peraltro per me - mi perdonerà, Presidente, la citazione personale - anche un esempio professionale, perché egli fu nominato - tutti lo ricorderanno - commissario liquidatore della Banca Banca privata finanziaria, una delle prime liquidazioni coatte amministrative disposte dalla Banca d'Italia, io in quell'epoca venivo incaricato di seguire una procedura di molta minore importanza e tuttavia per me l'avvocato Ambrosoli rappresentò un esempio.

la seconda volta, signor Presidente, quando l'ex ministro Diliberto, dopo aver scambiato la libertà della terrorista Silvia Baraldini con quella di tale Beneduce, che fu colui il quale fornì al mandante Sindona l'assassino materiale di Ambrosoli *(Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP)*, si recò all'aeroporto di Ciampino per assistere all'importazione, alla nazionalizzazione della terrorista Baraldini. Credo che in quel momento l'avvocato Ambrosoli fu ucciso per la seconda volta da un esponente di questa vostra maggioranza.

Questo è il Parlamento italiano, che ha il diritto e il dovere di legiferare sulle materie in cui intende legiferare

di gattopardiana memoria per cui tutto cambia affinché tutto rimanga uguale. Allora, senatoreD'Ambrosio, con buona pace, abbia rispetto del Parlamento, che può anche sbagliare

l'avvocato Ambrosoli credo sia un patrimonio di ricordo civile, professionale e umano

credo, senatore D'Ambrosio, che faremmo torto a tanti altri generosi operatori della giustizia e delle professioni

per motivi cruenti e assassini, noi non li ricordassimo, ma allora trasformeremmo quest'Aula in un ricordificio continuo di questo nostro triste passato! Io credo, senatore D'Ambrosio, che il tempo ha questa grande virtù, quella di non cancellare dalle nostre menti quelli che con noi più non sono, di ricordarli nei loro valori, ma di lasciarli anche in pace e

Mi è parso fuori misura per una persona come il senatore D'Ambrosio, normalmente così misurata, oltre che in quest'Aula anche fuori,

la sublimazione di un ricordo, fare attività di benevolenza, di circuizione quasi del mondo forense. Non credo, senatore D'Ambrosio,

intervengo per due questioni molto rapide. Ringrazio anzitutto il collega D'Ambrosio per il ricordo dell'avvocato Ambrosoli, al quale desidero unire il ricordo molto grato del Gruppo dell'UDC per quanto Ambrosoli ha rappresentato nel nostro Paese.

Allora, qualunque modifica di quel testo sarebbe una cosa diversa. Voglio che sia chiaro questo punto perché do per scontato che non sarà messo in votazione questo testo che abbiamo, ma qualcosa di diverso. E allora, se sarà messo in votazione qualcosa di diverso, non è ciò che ha detto il senatore Brutti adesso.

Detto questo, intervengo ora in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.200 2.200 che propone la soppressione dell'articolo 2. Intervengo per rispetto a lei, Presidente, perché lei questo ha disposto che sia, ma francamente lo faccio in una condizione che non è mutata rispetto a questa mattina, quando cioè il Presidente di turno, su mia sollecitazione, ha chiesto che fossero sospesi i lavori dell'Aula per giungere per giungere ad un chiarimento sulle parole con cui il ministro Mastella si era espresso con riferimento a uno dei punti centrali dell'articolo 2, di cui io propongo la soppressione e di cui l'Aula voterà quindi la soppressione o invece

L'articolo 2, di cui raccomando la soppressione, incide su più aspetti del disegno di legge che stiamo esaminando nel suo complesso. Uno di questi aspetti è quello che ho indicato illustrando gli emendamenti nel loro complesso, altro è invece quello su cui è intervenuto il senatore Brutti nel corso dell'illustrazione dell'emendamento che proprio poc'anzi ho indicato, quello della separazione delle funzioni.

che vorrebbe che il magistrato requirente non fosse mai separato nella propria carriera dal magistrato giudicante e che vi fosse unicità di carriera per tutti i magistrati. Il senatore Brutti ha, in tutta evidenza, legittimo diritto di pensarla come vuole; io sono, viceversa, di altra non assolutamente opposta opinione e credo di avere anch'io analogo diritto. Sulla questione della separazione delle carriere sono stati eretti due *totem*, uno dall'Associazione nazionale magistrati, che si è fieramente schierata contro tale separazione - e il senatore Brutti è fiancheggiatore di tale corrente di pensiero, come ho detto - l'altro dagli avvocati che, soprattutto in un certo periodo, in una certa epoca, si sono invece schierati assolutamente a favore

delle carriere, ma come deve essere individuata la figura del pubblico ministero, una volta che sia modificato l'assetto attuale. Più volte ho detto e ancora sostengo che il vero problema

discrezionalità dell'azione penale del nostro sistema; la vera questione è non mantenere il Paese isolato dall'Unione Europea, alla comunione dell'Europa rispetto ad una figura centrale per il funzionamento della legalità e perché sia assicurata la legalità dello Stato quale è quella del pubblico ministero. ministero. Il problema dei problemi, signor Presidente, è l'indipendenza o la non indipendenza del pubblico ministero. Su questa impostazione ho costruito una tesi,

e che su questo punto rischia davvero di trovarsi in futuro un Parlamento più libero e più coraggioso, che andrà ben oltre gli obiettivi conseguiti dalla riforma Castelli - di di cui oggi assistiamo allo smantellamento - con la separazione delle funzioni: una separazione seria, l'individuazione di due diversi mestieri, una separazione delle funzioni che fosse attuata anche attraverso strumenti surrettizi, qual è il divieto di rimanere

la cui sorte evidentemente non interessa a nessuno, nonché un rischio fortissimo di destabilizzazione organizzativa nei tribunali minori, che nel nostro Paese la prevalente maggioranza. Inoltre, nella puntuale applicazione di un emendamento come quello articolato dal senatore Brutti, cioè di quel modello che salva il *totem* ma distrugge il servizio e l'organizzazione, rischia davvero di non poter essere attuato e praticato. La raccomandazione che

vorrei molto rapidamente rispondere ai due interventi del collega Caruso. Sono un po' stupito del fatto che questo valoroso collega, per discutere e polemizzare sul merito di proposte che sono sul tappeto e che richiedono un confronto vero e serio, ricorra alla scorciatoia dell'insulto. È inutile dire che il proprio interlocutore è un ventriloquo, perché così si possono compiacere alcuni tifosi, ma non si aiuta il dibattito e non si raggiunge una conclusione che può essere soddisfacente per i tifosi, per i non tifosi e per il lavoro che dobbiamo svolgere in Parlamento. Parlamento. Ciò vale a rispondere ad un collega che apprezzo, ma al quale chiederei sommessamente un linguaggio che sia più adatto al nostro confronto parlamentare. In secondo luogo, non ho nessuna difficoltà a rispondere alle insistenti domande dei colleghi di centro-destra, i quali ci chiedono qual è il punto di ricaduta

ma poiché l'emendamento è mio ed è espressione della maggioranza, mi permetterà di dire come penso che si possa apportare una modifica lieve che aiuti il nostro lavoro e su cui l'intera maggioranza possa essere d'accordo. Chiedendo

- rappresenti la sconfitta clamorosa del Parlamento di fronte ad altre forze e ad altri poteri. Si farà la pace, certo, ma attraverso una resa ignominiosa.

è riunito un Comitato ristretto e questo emendamento non è mai uscito alla luce, neanche questa proposta. Sono state assunte decisioni diverse, con l'accordo del Governo e del relatore.

So che è un uomo d'onore e, di fronte al crollo di questo provvedimento, si sarebbe dimesso. A quel punto, non vedo come il Governo avrebbe potuto rimanere in piedi. Stiamo parlando di questo. Allora ci dovete dire attraverso quali artifici e ragionamenti, ma soprattutto attraverso quali pressioni, nascono determinati emendamenti. Infine, senatore Brutti,

piace. Al massimo può riformularlo, a giudizio della Presidenza. Quindi, non può modificare un bel nulla. Se vuole, lo può consegnare al Governo ed al relatore che possono presentare un emendamento, ma a quel punto chiediamo il tempo per presentare subemendamenti, cosa che sarebbe un dato assolutamente nuovo. È chiaro che finché non si dirime questo tema, noi stiamo in un certo modo aspettando Godot. Vogliamo capire esattamente di cosa stiamo parlando. Altrimenti assistiamo al senatore Brutti che prima dice

il collega Castelli si è ripetutamente rivolto a me e naturalmente ciò non può che farmi piacere e inorgoglirmi, nel senso che egli individua in me un interlocutore e anche un bersaglio. Bene così, questo è il confronto parlamentare: è anche battaglia e noi siamo pronti, caro collega Castelli, a sostenerla. Vorrei però per un momento accantonare i toni della battaglia e chiarire puntualmente qual è, a mio avviso, anche tenendo conto dell'intervento sincero e serio del collega D'Ambrosio, che ringrazio vivamente per le parole pronunziate, il possibile aggiustamento del mio emendamento 2.134 (testo 2), che rimane in piedi così com'è e che sottopongo all'attenzione dell'Aula, anche se fuori tempo perché ancora non siamo arrivati alla sua votazione. Comunque, non ho difficoltà a precisarlo fin da adesso, in modo che ciascun collega lo valuti attentamente. Prima però di passare a questo aggiustamento, che ha il consenso della maggioranza e che sottopongo ai colleghi, vorrei osservare che nel primo lungo periodo di questo emendamento c'è un refuso che vi prego di correggere. Signor Presidente,

da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario...». Nel punto in cui si dice: «da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale»,

comprendente più distretti ai magistrati che si muovono dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa nell'ambito del penale. Quindi, non avrebbe senso riproporre in relazione al passaggio dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni giudicanti civili. Si tratta pertanto di un puro refuso, che prego di correggere e che segnalo alla Presidenza. L'aggiunta

dell'ultimo periodo, cioè prima delle parole: «La destinazione alle funzioni giudicanti civili...», propongo di inserire la seguente breve frase: «In tutti i predetti casi

di trasferimento formulato in termini generali i magistrati che si spostano dalle funzioni giudicanti civili alle dalle funzioni giudicanti civili alle funzioni requirenti penali e, viceversa, dalle funzioni requirenti penali alle funzioni giudicanti civili. Nel caso però in cui si realizzi questo passaggio deve comunque esservi un mutamento di circondario, un trasferimento da un circondario all'altro. raccoglie le indicazioni e le critiche che erano state rivolte dal collega D'Ambrosio, che ringrazio per aver anticipato anticipato una possibile soluzione, che formulo in questi termini con questa breve frase che si aggiunge al testo dell'emendamento, che per il resto rimane uguale, e che sottopongo alla valutazione e al voto dei colleghi.

il mutamento che ha indicato il collega Brutti è sostanziale, perché introduce un divieto che lui localizza nell'ambito del circondario. Il mutamento sostanziale comporta la possibilità e la necessità di un termine per i subemendamenti. È fin troppo evidente che noi potremmo anche ipotizzare un impedimento che riguardi non il circondario ma il distretto e l'impossibilità di rientro nel circondario dove si sono svolte le funzioni di tipo diverso. La prego

contrario è la sospensione dei lavori dell'Aula. Stiamo lavorando con un dibattito il più largo possibile, credo che nel giro di un'ora si possano presentare subemendamenti alla modifica testé indicata dal senatore Brutti.

l'emendamento del senatore Brutti è una riformulazione che non comporta modifiche sostanziali per cui la Presidenza lo accetta come ammissibile, oppure è inammissibile e quindi non si possono presentare subemendamenti: *tertium non datur*.

Signor Presidente, quando prima ho dichiarato il voto sul mio emendamento soppressivo 2.200, non sarebbe stata la stessa cosa se l'emendamento fosse stato di altro tipo. Si mantiene o non si mantiene l'articolo 2. Avevo richiamato la sua attenzione proprio su questo fatto, su che cosa discutiamo, su che cosa vogliamo sopprimere o su che cosa vogliamo mantenere. L'emendamento presentato dal senatore Brutti non è cosa di poco conto;

allora che il senatore Brutti parlava per conto di un'accreditata Associazione di altissimi funzionari dello Stato, mi sembrava di non volere indicare un disvalore. Lui invece ha inteso che lo fosse. Prendo atto del fatto che sta modificando la propria prospettiva su questo

fosse giudicato non abbastanza quello che il Ministro e la maggioranza finora avevano fatto sotto dettatura di essa Associazione, ma fosse ritenuta necessaria questa ulteriore modifica, che, a posteriori rispetto al momento in cui lei ha disposto che io dichiarassi il voto, il senatore Brutti ha avuto la compiacenza di comunicare all'Aula. Signor Presidente, credo che la serietà e la ragionevolezza dei nostri lavori impongano due cose. Da un lato, ciò che ha chiesto il senatore Centaro. Gli emendamenti, signor Presidente, li facciamo noi (nel caso che mi riguarda, li faccio io), non sono appaltati ad altri; se sono in Aula, non posso stare a scrivere emendamenti. Si tratta di un punto centrale della questione. Credo che questo possa avvenire o adesso, come forse l'ordine dei lavori

che è stato poi sostituito da un emendamento aggiuntivo e che ora, di fatto, diventa un articolo aggiuntivo. Credo che tra la versione originale e questa non vi sia assoluta

Due più due fa quattro: questo dice l'emendamento; non dico una cosa del centro-destra, ma una cosa ovvia. Pertanto, lo mantengo, non lo ritiro e chiedo al relatore e al Governo di accettare l'emendamento perché è una proposta assolutamente banale e ovvia.

Mi sembra che la sostanza dell'emendamento sia recepita nel testo, perciò avevo detto che era superfluo; comunque, esprimo parere favorevole.

all'articolo 10, comma 16, scrivendo «con l'eccezione dei magistrati di cui al comma 16 dell'articolo 10». Questo serve a individuare come destinatari dell'esenzione dalla valutazione periodica i magistrati che hanno superato la settima valutazione di professionalità che, nel primo caso, sarebbero tutti, mentre, nel secondo caso, il procuratore generale presso la Cassazione e il presidente della Corte di cassazione, per evitare che si determini quella incompatibilità con la loro funzione di componenti, come membri di diritto, del Consiglio superiore della magistratura. Secondo me, la soluzione più *tranchant*, posto che stiamo parlando di magistrati che hanno già una carriera superiore a 30 anni, è quella di sopprimere le ultime quattro parole: «e, successivamente, ogni sei anni». È la soluzione più pulita e più precisa. Quindi, le chiedo di mettere questa nuova soluzione nuova soluzione in votazione.

prima che iniziasse la seduta di oggi pomeriggio si è avvicinato e mi ha detto: «Guarda che ninnillo vuol dire guaglioncello, in napoletano», e mi ha precisato che quel personaggio che io avevo evocato come protagonista di «Natale in casa Cupiello», nella realtà era un protagonista di «Miseria e nobiltà».

Presidente, ho un problema. Ricordo una pubblicità in cui c'era un signore, vestito con una sahariana, che girava tra le piante e controllando gli ananas diceva: «Questo sì, questo no». Nel dubbio che gli ananas, cioè gli emendamenti, di mia produzione fossero tutti acerbi, ho cercato di correggere il primo che sarebbe venuto all'attenzione del Senato, che mi sembrava non dico il più maturo, ma quello che poteva maturare più in fretta.

Secondo il testo,

l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove». Questo ha una sua logica, perché se nella valutazione di professionalità il valutante dovesse scendere sul piano di come sono state interpretate le norme di diritto ovvero di come è stato valutato il fatto vi sarebbe oggettivamente una lesione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Quello che crea problemi, e che io provo ad emendare, è l'inciso «in nessun caso», in quanto si prevede che qualunque sia l'errore commesso dai magistrati nell'interpretazione delle norme e nella valutazione del fatto non può essere considerato quell'errore ai fini della valutazione della professionalità del magistrato, il che peraltro appare strano se si considera che tra le fattispecie disciplinari, e cioè dei procedimenti disciplinari che possono essere svolti a carico dei magistrati, vi è, per l'appunto, l'errore macroscopico nell'interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto

il magistrato tizio subisce un procedimento disciplinare perché, ad esempio, ha emesso una ordinanza cautelare con restrizione in carcere al di fuori dei casi consentiti, perciò stesso subirebbe un procedimento disciplinare e, per ipotesi, la sanzione disciplinare conseguente, ma questo errore macroscopico accertato in sede disciplinare non potrebbe avere rilevanza sotto il profilo della valutazione della professionalità, essendovi scritto in questa norma «in nessuno caso». Allora, si chiede semplicemente all'Aula - ed è questa la ragione per cui non capisco il no per cui non capisco il no - di concordare la normativa generale con la normativa disciplinare e prevedere che quando si valuta il magistrato non è possibile interessarsi della interpretazione delle norme o della valutazione del fatto, a meno che

considerata foriera di errori. È la prova provata che il testo è stato scritto dalla magistratura, perché nessun parlamentare indipendente credo si sarebbe mai sognato di formulare una norma del genere. Oggi con questa norma viene sancita l'infallibilità del magistrato, che non sarà più soggetto solo alla legge, come prevede la Costituzione, ma sarà *legibus solutus*: questo è il dato.

Ebbene, se passa questa norma, è del tutto evidente che non ci potrà mai essere alcun provvedimento disciplinare che possa in qualche modo interloquire o interferire con una sentenza, qualunque essa sia, anche la più abnorme.

da una corporazione. Tra l'altro, colleghi, approfitto per anticiparvi una questione che non è mai emersa: già che c'erano, si sono anche aumentati lo stipendio, giusto per capirci; già che stavano scrivendo, perché non dare un ritocchino allo stipendio di qualche magistrato? L'occasione era troppo ghiotta. Poi siamo noi politici ad essere tacciati per i costi della politica, eccetera, eccetera, eccetera. *(Applausi

comma 2, sulla valutazione di professionalità prevede che tale valutazione non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, e così via. Tale norma molto opportunamente ci è stata suggerita

Credo che aggiungere «salvo in caso di errore macroscopico» sia improprio, perché tutto sommato l'errore macroscopico, seppure avrà una sua refluenza disciplinare, sarà poi giudicato nella valutazione di professionalità. Credo che, per la valutazione di professionalità, l'esame delle prove e dei fatti debba essere lasciato così com'è, anche perché

Hanno votato tutti?

Presidente, per evitare quella che lei chiama

Questa situazione è bilaterale e alla fine è ingovernabile anche per chi la determina, perché la risposta può travolgere anche la scorrettezza dell'altro. Senatori, posso chiedervi di restare ai vostri posti? Siamo una scolaresca

è contemplato, in queste fasi così eccitate, che lei nomini un garante dell'ordine? Io avevo pensato al senatore Garraffa, quel ragazzo con i baffi che è così garbato e gentile. Possiamo nominare Garraffa garante di tutti.

legittima aspirazione di ben figurare nel corso della carriera e di essere ottemperante ad uno dei parametri altrove stabiliti in sede di Consiglio superiore della magistratura)

coscienza e secondo conoscenza. Il rimedio deve essere endoprocessuale: se il magistrato sbaglia, come pure capita, occorre che il rimedio sia trovato all'interno del sistema e con il sistema. Troppo diverse sono le attribuzioni da magistrato a magistrato. Le sentenze, signor Presidente, non sono bistecche (con tutto rispetto per la professione del macellaio) che possono essere serialmente affettate, non tutti i processi sono uguali: avere la presunzione, la pretesa di stabilire uno standard che disciplini e governi l'attività del magistrato e a a cui sia subordinata la possibilità e, ripeto, l'aspettativa legittima di una carriera ordinata e virtuosa, non è cosa opportuna. Per questo chiedo sia soppressa questa previsione, come ripeto e torno a dire, ovunque essa ricorra. Chiedo, inoltre, che il relatore e il Governo riconsiderino il loro parere al riguardo.

che gli addetti ai lavori conoscono molto bene. Qual è stato uno dei problemi gravissimi che ha sempre avuto

dell'anno giudiziario 2006), il sistema è degenerato e gli incarichi direttivi sono sempre stati affidati attraverso una precisa lottizzazione, dominata dalle correnti che collocano i loro uomini nel Consiglio superiore della magistratura.

istituto forse complicato (può darsi, è una critica che può essere accettata), ma era evidente che bisognava introdurre elementi oggettivi. Cosa fa questo provvedimento, che interviene non soltanto sull'affidamento degli incarichi direttivi, ma addirittura sulla professionalità del magistrato con sanzioni che possono arrivare persino a mettere in mezzo alla strada il magistrato stesso?

quando si trattò di nominare il sostituto del procuratore capo Cordova, che venne spostato da Napoli con un provvedimento di natura eccezionale per incompatibilità ambientale; ciò avvenne con la motivazione

Siamo noi che difendiamo i magistrati, non voi; è questo il dato che deve emergere da questo Consesso e dalla nostra discussione. In questo momento siamo noi che stiamo cercando di difendere l'autonomia e l'indipendenza del magistrato contro lo strapotere delle correnti.

qualcosa che, per la verità, non ho mai sentito chiedere nel corso della mia militanza parlamentare e di cui, tuttavia, avverto la necessità. Più volte ho potuto constatare che i pareri che la Commissione bilancio esprime sui provvedimenti che esaminiamo sono simili alle parole di Zarathustra: quelle sono e quelle devono essere, senza alcuna motivazione e senza alcuna spiegazione. Nel caso del provvedimento che stiamo esaminando, ero e continuo ad essere della convinzione che i pareri resi dalla Commissione bilancio

previsioni contenute nel testo e poco importa se alcune di tali previsioni sono destinate - perché non è detto che obbligatoriamente lo siano ad essere stralciate. Quello che le chiedo, signor Presidente, è, in particolare, di poter acquisire alla documentazione fornita ai colleghi dell'Aula il della seduta della Commissione bilancio in cui è stato esaminato con una conclusione negativa, rafforzata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3, comma 11, capoverso 17-*ter*,

Castelli ha ragione, però, io provo ad argomentare i miei emendamenti perché ricordo che nella scorsa legislatura, nonostante vi fosse un fortissimo divario tra maggioranza e minoranza, almeno nelle materie in cui pensavo di avere un minimo di competenza, ho sempre ascoltato i ragionamenti dei colleghi e talvolta mi è capitato, condividendoli, di votare secondo la mia coscienza e non secondo il dito che mi veniva mostrato dal comitato dei nove, Questo emendamento, a mio modestissimo avviso, è tutto in favore dei magistrati e adesso con calma vi spiego le ragioni. I senatori Massimo Brutti, Buccico e Ziccone sono stati al Consiglio superiore della magistratura e vi potranno - credo - testimoniare quante denunce anonime o pseudoanonime (ove per pseudoanonime si intendono quelle denunce che trovano una firma, anche se poi quella firma e quell'indirizzo appartengono a persona diversa da quella che ha praticamente scritto la denuncia) arrivano arrivano al Consiglio stesso ogniqualvolta si tratti di conferire un incarico direttivo, semidirettivo o addirittura un trasferimento.

sono comunque oggetto di un cicaleccio nell'ambito dei corridoi. Nella norma in questione si dice sostanzialmente che il capo dell'ufficio, nel rilasciare il parere per la valutazione del magistrato, deve tenere conto delle segnalazioni su fatti specifici provenienti da terzi; il che equivale a dire che in quel momento il capo dell'ufficio sarà molto probabilmente destinatario di una serie di denunce, firmate da Ferruccio Saro o da Nitto Palma o da Emiddio Novi, oppure - se mi consentono, così facciamo un esempio *bipartisan* - da Massimo Brutti o da Gerardo D'Ambrosio, nessuno dei quali nella realtà è autore di quella denuncia, ma sono tutte e cinque persone esistenti con tali denunce si individua un fatto specifico - vero o falso che sia poco importa - a carico di un magistrato. Siccome il capo dell'ufficio non ha il potere di compiere gli accertamenti su quella denuncia - è chiaro che, se quegli accertamenti hanno una valenza diversa, l'organo competente è altro terrà o non terrà in considerazione quelle denunce, immagino io, secondo il gradimento che ha nei confronti del magistrato da valutare. Il senatore Calvi, se mi presta un secondo di attenzione tra una telefonata e l'altra, ricorderà quando, ai tempi della procura di Roma (non era esattamente la procura di Roma), un capo dell'ufficio chiamava il magistrato e diceva: «Sai, mi è arrivata una cosa nel cassetto, ma siccome sei mio amico la lascio lì». Parliamo di molti e molti anni fa. Bene, voi cercate sostanzialmente di ripetere una situazione del genere, cioè di ancorare, o meglio, di dare al capo dell'ufficio la possibilità di esprimere una valutazione positiva o negativa sostanzialmente sul nulla, perché nulla sono le segnalazioni provenienti da terzi che non hanno ricevuto un approfondimento di carattere accertativo. Quindi, come vedete, questo è un emendamento a favore del magistrato. Così come, mi rendo conto della diversità del termine, però, scusatemi, io propongo che invece delle segnalazioni del consiglio dell'ordine vi sia un parere da del consiglio dell'ordine. Non riesco a comprendere. Capisco che la segnalazione è qualcosa che pesa di meno per i magistrati, ma siccome in termini istituzionali l'interloquire tra un organo e un altro si chiama parere mi sembrerebbe più corretto parlare di parere.

e cioè dei dati che sono a sua conoscenza in base all'attività lavorativa del magistrato, di un parere che arriva da un organo pubblico, perché pubblico è il consiglio dell'ordine degli avvocati, e di evitare che tale valutazione possa essere in un modo

Hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione.

Signor Presidente, il testo che propongo è nella sostanza uguale a quello già previsto dal disegno di legge, quindi di per sé l'emendamento potrebbe essere ritirato perché pletorico.

che ai commi 11 e 13, anche al comma 7, che è stato evidentemente dimenticato e in cui pure è prevista un'ipotesi di audizione del magistrato e dunque del suo difensore.

Presidente, questo compito meramente esecutivo del Ministro della giustizia è esteticamente imbarazzante. Il Ministro prende atto delle determinazioni sulle valutazioni di professionalità e dà corso al decreto. Attraverso l'emendamento gli si consente un'eventuale ricognizione. A volte le valutazioni possono anche confliggere con quanto è notorio e il Ministro può quindi adottare delle determinazioni diverse. Ritengo che sotto questo profilo meriti attenzione la proposta e confido nel voto favorevole dell'Aula.

Hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione.

Dichiaro aperta la votazione. *(Segue la votazione).* Hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione.

credo che anche questo sia un emendamento cha va sostanzialmente nel senso voluto addirittura dall'Associazione nazionale magistrati.

i posti di consigliere di Cassazione, cioè i posti di legittimità, per un 10 per cento sono riservati ai magistrati che non hanno l'anzianità necessaria per ottenere le funzioni di legittimità normalmente: sostanzialmente quelli che hanno maturato il secondo o il terzo passaggio di anzianità. Orbene, ricordo che una volta arrivò un magistrato a fare il procuratore della Repubblica di Roma; era bravissimo e il collega Sica, nel dare atto della bravura di questo magistrato, disse: «Ma siete davvero sicuri che chi conosce a memoria l'enciclopedia dello sci sa sciare?». Con questo cosa voglio dire? Che cosa pensate voi che sia un magistrato?

Davvero voi ritenete che quello che importa più di tutto per un magistrato, tanto da conferirgli con un anticipo di svariati anni le funzioni di legittimità, semplicemente, oltre che dall'aver svolto in maniera egregia il proprio lavoro, dall'aver scritto qualche articolo scientifico? Vede, senatore Castelli, rispetto alla sua riforma, vi è una differenza sostanziale. Nella riforma Castelli l'anticipazione di carriera si ancorava a un concorso per esami, cioè ad un dato oggettivo, ad una serie di compiti scritti che venivano valutati in maniera omogenea dalla commissione.

se conferire a Tizio, a Caio o a Sempronio le funzioni di legittimità con diversi anni di anticipo rispetto al momento in cui questi signori avrebbero potuto ottenerle secondo anzianità. Bene, vorrei dire ai signori del centro-destra e anche a quelli del centro-sinistra: fate attenzione, perché voi in questo modo consentite al Consiglio superiore della magistratura di prefigurare con largo anticipo le carriere di taluni magistrati e di mettere le basi per conferire successivamente a questi magistrati gli incarichi direttivi di maggiore prestigio. [**Presidenza del vice presidente è quella di evitare che l'inquinamento correntizio che si sviluppa attraverso il Consiglio superiore della magistratura possa continuare ad incidere così pesantemente sull'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, voi questa norma, a mio avviso, la dovete sopprimere; e la dovete sopprimere - ripeto - perché è una norma profondamente ingiusta e che lascia, come al solito, alle camarille associative in sede consiliare la possibilità di prefigurare grandi carriere in favore dei magistrati amici.

Prego i colleghi di prendere posto, per favore. Dietro

prego, senatore l'aggiunta solo a «l'aver prestato servizio in sedi disagiate» e quindi considerando estromessa dall'emendamento la frase «l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie giudiziarie ». Si sta qui parlando dei criteri con cui devono essere valutati i magistrati per il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive.

che hanno una certa anzianità e che, invece di restarsene in centri di tutto comodo, vanno a svolgere il loro lavoro in centri come Locri, Reggio Calabria, Palermo, Caltanissetta, Catania,

mi dovete spiegare la ragione - e su questo di nuovo il senatore Buccico potrebbe essermi testimone - per la quale a Locri non ci sono magistrati esperti, perché in centri di assoluta invadenza criminale non vi sono magistrati esperti. Qual è, scusate, la ragione per la quale un magistrato bravo, un magistrato esperto dovrebbe andare a Locri senza poi averne un ritorno corretto sotto il profilo della carriera? Senatore Brutti, credo che lei sorrida perché evidentemente condivide il mio dire, ma nell'eventualità in cui il suo sorriso non dovesse essere di condivisione ma di altro, la prego allora di spiegarmi davvero la ragione per la quale i magistrati esperti e di grande capacità in questi centri non ci vanno mai. Vede, senatore Brutti, ho un ricordo: ho avuto le funzioni in magistratura nel maggio 1978, una epoca in cui per rientrare a Roma ci volevano otto, nove, dieci anni: ebbene, sono rientrato a Roma nel settembre 1979, perché i tanti, troppi morti che vennero fatti dalle Brigate rosse e dall'eversione di destra avevano, chissà perché, svuotato la procura di Roma. Io ebbi la possibilità di rientrarvi dopo un anno, purtroppo, o fortunatamente, sono stato impegnato in reati di terrorismo e di criminalità organizzata, bene, senatore Massimo Brutti, non lo desideravo all'epoca, però davvero la prego di credermi che nessun vantaggio questo ha costituito per la mia carriera. Allora, smettetela di essere ipocriti, quando in quei centri pericolosi troverete solo ragazzini che ci vanno, non perché ci desiderano andare, ma perché probabilmente sono gli ultimi in graduatoria e quello è l'unico posto che a loro compete, con grave detrimento per l'efficienza dell'azione repressiva dello Stato e, scusatemi tanto, anche per la stessa immagine che lo Stato consegna della magistratura al Paese.

Abbiamo previsto che chi svolge le sue funzioni per cinque anni in una sede disagiata, poi avrà la precedenza assoluta su tutti nel trasferimento.

a Gela e che poi erano rimasti intrappolati lì a seguito di una modifica della legge, erano rimasti lì prigionieri dopo aver scelto quella sede disagiata credendo di poter usufruire del premio meritato. Quindi, abbiamo appieno appieno risposto all'esigenza di questi magistrati, per cui vi chiedo di respingere l'emendamento, perché già abbiamo provveduto a parte.

La sede disagiata è determinata dalla vacanza del posto, per cui in definitiva in queste sedi disagiate non vanno i magistrati migliori, migliori, ma quelli meno esperti, che si trovano con un carico di lavoro spaventoso ad affrontare problemi che non hanno mai affrontato durante la loro vita; sono i magistrati più giovani, che avrebbero bisogno di maturare altrove le loro esperienze. Con questo emendamento, invece, secondo me, il senatore Palma pone un problema serio e concreto. Se andiamo ad incentivare l'esperienza e l'orgoglio dei magistrati più preparati, in quelle sedi effettivamente disagiate (dove deve mutare il meccanismo della sede disagiata come scelta operativa per i magistrati) andremo a creare effettivamente una barriera contro la criminalità organizzata. L'ottica attraverso cui viene proposto questo emendamento è quindi da quella che pone il senatore Di Lello. Mi sembra si tratti di un emendamento di civiltà, che pone per la prima volta una gerarchia di valori sul piano delle scelte da parte dei magistrati. Se vogliamo invece continuare a mandare negli avamposti della criminalità (quelli che sono stati citati dal collega Di Lello: Caltanissetta, Gela, Locri) i magistrati meno esperti, i ragazzini, coloro che vengono sopraffatti poi dalla criminalità organizzata, continuiamo a chiudere gli occhi e ad operare queste scelte di retroguardia.

Palma. Posso dare la parola per un minuto per un puro fatto di cortesia parlamentare, ma non di più. La prego, senatore Centaro, si attenga al rispetto Presidente, la ringrazio per il tempo che mi è stato accordato. Intervengo giusto per far notare che le argomentazioni del collega Di Lello valgono per il primo trasferimento, ma per il conferimento di uffici direttivi e la valutazione complessiva di una carriera è importante verificare la laboriosità, ma anche il sacrificio che tanti magistrati hanno volutamente ed espressamente fatto trasferendosi in quelle sedi. Si tratta quindi di cosa diversa rispetto a ciò che ha argomentato il collega Di Lello.

Voteremo a favore di questo emendamento. Approfitto della parola per segnalare all'Aula una questione legata alle argomentazioni che hanno testé svolto così efficacemente sia il senatore Palma che il senatore Buccico, per denunciare come sia caduto molto in basso l'impegno in questa legislatura contro la criminalità organizzata. Mi riferisco a come è nata la Commissione di una Commissione che, per volontà della maggioranza, è nata già morta, asfittica. Pensate che deve fare i conti con un bilancio globale di 300.000 euro all'anno, con il quale devono essere pagate tutte le trasferte,

di 100 miliardi di euro e noi la combattiamo con 300.000 euro all'anno. Questo è quello che ha fatto questa maggioranza in termini di lotta alla criminalità organizzata. Vi è di più: è stato nominato come Presidente un parlamentare di prima nomina, quindi evidentemente inesperto delle questioni. Non possono nominare consulenti perché non hanno i soldi per pagarli. Non possono andare a fare le loro indagini *in* *loco* perché non ci sono i soldi per pagare le trasferte. Insomma, è stata creata una creata una Commissione già morta. Credo che anche la bocciatura di questo emendamento vada in questa direzione: nella direzione per la quale la lotta alla criminalità organizzata questa maggioranza la fa molto a parole ma molto poco nei fatti.

A quello che ha detto il senatore Di Lello va aggiunta una considerazione: il solo fatto di aver prestato servizio in una sede disagiata non può essere di per sé titolo preferenziale per un incarico direttivo perché purtroppo in tante sedi disagiate del Sud d'Italia (della Calabria piuttosto che della Basilicata o della Sicilia) prestano servizio magistrati con risultati non eclatanti, per usare un eufemismo. Se si vuole dunque tener conto di questo dato, bisogna quanto meno dire: «l'aver svolto l'attività in sedi disagiate, con risultati positivi nella lotta contro la criminalità organizzata». conoscendo onestamente un po' il quadro della realtà meridionale, non mi sentirei di dare una medaglietta a tutti i magistrati che in questo momento prestano servizio nelle sedi disagiate.

Signor Presidente, ho ascoltato il suggerimento del collega Salvi, ma non è per me convincente, perchè si sovrappone alla valutazione della professionalità del magistrato una logica del risultato. Noi siamo, invece, alla valutazione della professionalità, che può anche, in condizioni avverse, non produrre risultati nella lotta contro la criminalità organizzata o produrne meno di quanti quel magistrato volenteroso vorrebbe. Faccio però una proposta, dal momento

che non faccia riferimento alla logica del risultato, ma che sia tale da qualificare quella permanenza nella sede disagiata, che riteniamo degna di considerazione positiva, ai fini della valutazione di professionalità.

al di là della laconicità dei numeri, è bene che l'Aula faccia attenzione a quali sono le funzioni previste dai commi 9, 10 e 11 funzioni direttive giudicanti di primo grado, quelle cioè di presidente del tribunale; presidente di tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città particolarmente ampie; le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, cioè quelle di presidente di corte d'appello. d'appello. Ritengo sia doveroso, prima di conferire incarichi di questa levatura, sottoporre a ricognizione attenta i requisiti di coloro che andranno ad occupare queste posizioni così importanti. Francamente non vedo perché questi requisiti debbano essere limitati soltanto a coloro che diventeranno poi primo presidente di Cassazione o procuratore generale di Cassazione. Noi ci confrontiamo sistematicamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, con problemi che nascono - sempre per usare un eufemismo per attitudini non verificate di magistrati che governano uffici periferici con posizioni apicali, città provinciali cui i capi degli uffici non hanno requisiti particolari e da quelle città poi partono devastanti pregiudizi per la collettività. Ora, francamente, non vedo la ragione per la quale chi vada ad occupare quella posizione non debba sottoporsi a una verifica più rigorosa, più puntuale e penetrante, le sue attribuzioni ed attitudini non debbano essere controllate con tutte le attenzioni possibili da parte del Consiglio superiore della magistratura. Veramente, escludere capi di uffici importanti da considerazioni e valutazioni che sono perfettamente conferenti rispetto alla posizione che andranno ad occupare mi sembra assolutamente riduttivo. Non ci possiamo lamentare di ciò che accade. Il Parlamento ha una grande responsabilità in questo momento; anche se non colgo un'attenzione particolare,

che questo emendamento, di cui raccomando l'approvazione e su cui il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore, venga riformulato. Del resto, credo di avere qualche giustificazione per il fatto che, come lei sa, signor Presidente, questo testo estremamente complesso e complicato è stato affidato alla disponibilità dei senatori con grande ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione degli emendamenti. Pertanto, anche negli emendamenti stessi, almeno nei miei, si hanno delle aporie che vanno rimediate.

in cui si passano in rassegna i commi da 12 a 16 dell'articolo 10, cioè tutte le funzioni direttive, per stabilire quando le stesse possono essere ricoperte. Per esempio, il comma 7 afferma: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità». Il magistrato deve quindi avere venti anni di carriera. La seconda parte è rappresentata dai commi

con essa si stabiliscono invece quali sono i criteri in relazione a ciascuna delle funzioni direttive alle quali il magistrato può legittimamente aspirare. Ebbene, nella riscrittura del testo, dopo il passaggio in Commissione, come lei signor Presidente può vedere, sono saltati i riferimenti ai commi 12 e 13, nel senso che al comma 10 si fa al comma 10 si fa riferimento ai commi 7,8,9, 10 e 11 dell'articolo 10, mentre al comma 11 si fa riferimento ai commi 14, 15 e 16; i commi 12 e 13 invece sono scomparsi,

richiesti vi deve essere quello della frequenza dei corsi anche antecedenti all'entrata in magistratura, ma deve essere una frequenza coronata da un esito positivo, da una certificazione di qualsiasi tipo - e questo mi sembra

perché, fra l'altro, si raccorda ad una previsione contenuta nel testo proposto all'Aula dalla Commissione, con riferimento all'attività della Scuola superiore della magistratura che prevede la necessità che in caso di conferimento di funzioni direttive o in caso di mutamento di funzioni vi siano dei corsi di formazione al riguardo presso la stessa scuola la quale a sua volta invierà una relazione sulla frequentazione del corso da parte del magistrato. L'indicazione dell'esito positivo fa riferimento ad una relazione che comunque verrà inviata, e logica vuole che evidentemente ci si riferisca ad una relazione che dia esito positivo. Se noi lasciamo semplicemente l'indicazione della frequenza di un corso di formazione ai fini della valutazione degli uffici direttivi, ci riferiamo ci riferiamo ad un dato obiettivo dimenticando che tale dato obiettivo sarà comunque accompagnato da una relazione, ancorché non considerabile valutazione, in quanto le valutazioni sui magistrati, come è noto, possono essere svolte solo dal Consiglio superiore della magistratura. Ciò premesso, questa aggiunta a me pare assolutamente in linea e in sintonia con norma già approvata dalla Commissione e proposta all'Aula.

e riguarda la riserva di giovani magistrati che dovrebbero, saltando alcuni passaggi, adire alle funzioni di legittimità. legittimità. Colleghi, vi è una questione che i magistrati difendono a denti stretti e a spada tratta, come se fosse un loro bene irrinunciabile e che a me, *absit iniuria verbis*, sembra veramente triste. Che cosa accade oggi nella magistratura? I magistrati fanno carriera solo ed esclusivamente in funzione dell'età. Mano a mano che l'età avanza, avanzano in carriera. Questo a me sembra di una tristezza incredibile. Pensate: è tolta ogni speranza! Un giovane brillante non può pensare di fare carriera rapidamente perché più bravo degli altri, ma è costretto ad aspettare che si incanutisca, si ingrigisca,

in maniera incredibile dai magistrati perché, nella mia vita non ho mai accettato una situazione del genere. Ho sempre cercato di nuotare nel mare magno del mercato, cercando di acquisire, più o meno modestamente, quei meriti che ritenevo potessi acquisire. Abbiamo cercato di portare questa mentalità anche all'interno della magistratura, non per creare dei valori di mercato o una concorrenza, ma per garantire a qualche giovane una speranza in più. Allora abbiamo introdotto una norma che garantiva la possibilità a giovani magistrati, attraverso un concorso, di poter adire immediatamente alle funzioni di legittimità, cioè in Cassazione. Questa norma è passata con la grande opposizione dell'Associazione nazionale magistrati, ma ne rimane qualche eco in questa legge. Evidentemente la *ratio* era considerata condivisibile, visto che anche in questo caso

alleverà i suoi pulcini migliori. Questo è già un caso che non è più troppo fisiologico. Nel terzo caso, siamo in Italia, magari il figlio di qualcuno che nel CSM è potente farà carriera più rapidamente degli altri. Questo è il quadretto che anche in questo caso

(quindi, non mi si venga a dire che io obbligo ai concorsifici), ma sarebbe soltanto facoltativo per quei giovani ambiziosi che si ritengono più capaci di andare in Cassazione.

**Il Senato non approva.**

in un convegno sull'ordinamento giudiziario il consigliere Nello Rossi, esponente di punta di Magistratura democratica, affermò che il Consiglio superiore della magistratura aveva fallito il suo compito sotto il profilo della selezione dei magistrati. dei magistrati. Affermava che con riferimento alla scelta dei titolari degli incarichi semidirettivi o direttivi il Consiglio superiore aveva sbagliato, forse perché troppo succube delle pressioni e delle correnti. Badate bene che non lo dico io, lo diceva il consigliere Rossi e se, per ipotesi, doveste avete dei dubbi, dato che lo sto riferendo io, troverete il testo dell'intervento su «Cassazione penale» del 2003. Nello stesso testo troverete un'affermazione del presidente Marvulli, all'epoca presidente della Cassazione, il quale confermava che nella scelta dei capi degli uffici il Consiglio superiore della magistratura non aveva dato gran prova di sé e che si doveva immaginare un sistema diverso.

che il Consiglio superiore istituisse una commissione che procedesse alla verifica dei titoli presentati dai vari magistrati ed esprimesse una proposta motivata, che il Consiglio superiore accogliesse, ovvero, nell'eventualità in cui volesse discostarsene, respingesse con parere contrario. Questo è esattamente quanto, con riferimento alle funzioni di legittimità, è contenuto nel testo di legge varato dalla Commissione. Per il conferimento delle funzioni di legittimità il Consiglio superiore deve seguire il parere espresso da una commissione e per discostarsene deve farlo con parere motivato. A me non pare che gli incarichi direttivi e semidirettivi, ossia i capi degli uffici, abbiano responsabilità minori rispetto alle responsabilità di un consigliere di Cassazione. Né mi pare che il Consiglio superiore, che attraverso questa norma viene indicato come non particolarmente idoneo a valutare i titoli scientifici dei magistrati, abbia la competenza per verificare le capacità organizzative di direzione dei magistrati, considerando che nella stragrande maggioranza, con riferimento alla componente togata, è composto di magistrati di scarso livello di anzianità.

votando no consentirete che continui la prassi al Consiglio superiore della magistratura del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi non a chi realmente li merita, bensì secondo spartizioni correntizie. Consentirete che incarichi direttivi e semidirettivi rimangano fermi per sei mesi, per un anno, per un anno e sei mesi finché non si liberino analoghi incarichi direttivi in modo da poter arrivare a una spartizione tra le varie correnti. Tale spartizione - si badi bene - non va a premiare necessariamente i magistrati più bravi e più preparati di quelle correnti, ma i magistrati correnti, ma i magistrati associativamente più omogenei. Tutto qui. Quando un ufficio è diretto da un capo dell'ufficio o è semidiretto da un semicapo dell'ufficio non all'altezza,

quando vi troverete di fronte a capi degli uffici non all'altezza. Mi rendo però conto che per l'attuale composizione del Consiglio superiore è per voi conveniente che questa norma non venga approvata, perché attraverso i giochi da talune correnti e della vostra politica sarete in grado di presidiare il territorio. Chiedo scusa, ma è stato un *lapsus* dovuto alla mia vecchia professione. Non intendevo dire di presidiare e di controllare il territorio, ma di presidiare e controllare, attraverso la vostra *longa manus*, gli uffici giudiziari, con buona pace dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Sembra che l'intervento del collega Palma abbia toccato la sostanza e il nocciolo della questione. È vero che l'Associazione nazionale magistrati avrebbe forse preferito una norma che disciplinasse l'ordinamento in modo meno che entrasse meno nelle pieghe della carriera e dell'operato dei magistrati e della loro valutazione.

Perché questa necessità di trovare numeri e artifizi, per poi vanificare tutto questo? questo? Discutendo all'interno del mio Gruppo, io sostenevo la tesi che forse il mio collega Castelli era fino troppo buono e morbido nell'affrontare le garanzie

non positivo (o negativo) che avrebbe bloccato la loro carriera fino al punto di poterli espellere dall'ordinamento giudiziario. E quale sarà il metro? È probabile che, se il CSM è quello che abbiamo conosciuto (lottizzato, politicizzato e fortemente caratterizzato da una connotazione politica attuale), tutti i magistrati che sono fuori da quell'area

in primo luogo dalla conoscenza del costume e della cultura del posto. Perché non si è mai introdotto un criterio localistico di selezione dei magistrati?

In Sicilia non si amministrava la giustizia come in Piemonte, in Sardegna non si amministrava come nel Lazio; il codice barbaricino lo si faceva vigere solo per la Sardegna, mentre il delitto d'onore era considerato un'attenuante soltanto in Sicilia, non nelle altre parti del territorio. Bisognava avere coscienza della cultura

Presidente, rimango un po' sbalordito dal contenuto dell'emendamento 2.123 del senatore Palma, per la parte che concerne la sostituzione, così come viene proposta.

dall'opposizione. L'emendamento propone, per il conferimento di determinate funzioni elevate di cui dirò tra poco, di eliminare alcuni requisiti, che invece io ritengo fondamentali. Tutta la parte dell'articolo e del comma per la quale viene chiesta una sostituzione concerne requisiti importanti che abbiamo valutato ampiamente all'interno del comitato ristretto della Commissione giustizia e nella Commissione plenaria stessa. Si tratta, in particolare, di una valutazione che deve essere effettuata in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, anche per quanto riguarda il conferimento di funzioni molto elevate.

alla valutazione che deve effettuare l'apposita commissione del Consiglio superiore della magistratura sulla capacità scientifica del magistrato che deve essere nominato a funzioni elevate e sulla capacità di analizzare nel dettaglio le norme; si tratta di requisiti che riteniamo fondamentali. Infatti, così come verrebbe tagliata la norma, cioè come verrebbe tagliato questo comma, porrebbero problemi di criteri e di requisiti per la valutazione del magistrato stesso perché quell'apposita commissione del Consiglio superiore della magistratura potrebbe soltanto far riferimento a requisiti generici precedenti, ma non ad una valutazione specifica, così come è stata indicata dall'articolato che viene proposto dalla Commissione giustizia. C'è, inoltre, un'altra considerazione che va effettuata. Dopo una lunga discussione da parte della Commissione giustizia, eravamo giunti all'individuazione delle funzioni giudicanti e requirenti per le quali era necessario procedere con questa apposita commissione secondo una procedura particolare e con la richiesta di requisiti particolari, tant'è vero che, appunto dopo quell'approfondita analisi della Commissione giustizia, avevamo individuato la necessità di richiedere quegli specifici requisiti solamente in riferimento alle elevate funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, sempre di questo decreto legislativo. Le funzioni elevate di cui al comma 5 sono essenzialmente le funzioni giudicanti di legittimità (che sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione) e, inoltre, le funzioni requirenti di legittimità, che sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. Mi giunge, invece, incomprensibile per altri versi, dopo le valutazioni che avevamo già effettuato, questo allargamento, oltre che al comma 5, anche ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo del decreto in questione. Il riferimento a queste altre funzioni, infatti, mal si confà rispetto all'impostazione della norma,

di cui ai commi 9, 10, 11 e 12, vediamo che si tratta di funzioni tutt'affatto diverse rispetto a quelle che hanno determinato le scelta della Commissione giustizia. Le funzioni di cui al comma 9 sono le funzioni direttive giudicanti di primo grado e quindi, in particolare, sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, mentre le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario come quelle di procuratore della Repubblica per il tribunale dei minorenni. Una situazione analoga e delle considerazioni analoghe devono essere effettuate per quanto riguarda il comma 10 di questo articolo. Si parla qui di funzioni direttive giudicanti elevate, che sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente dei tribunali di sorveglianza, facendo però caso che si tratta di uffici particolari; non di tribunali ordinari quindi, ma di tribunali che hanno una competenza specifica all'interno del distretto. Tali funzioni fanno riferimento ai maggiori tribunali che che sono dislocati in tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda, invece, le corrispondenti funzioni direttive requirenti elevate di primo grado ci si riferisce alle funzioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di queste specifiche e speciali città che sono le città principali ubicate in tutto il territorio nazionale. Anche il riferimento al comma 11 ci rende contezza della scelta ponderata e adeguata della Commissione giustizia perché ci si riferisce alle funzioni direttive giudicanti di secondo grado e queste sono in maniera palese e chiara le funzioni del presidente di Corte d'appello; così come le corrispondenti funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle del procuratore generale presso la Corte d'appello. L'ultimo comma che si vorrebbe inserire con l'emendamento 2.123, del senatore Palma, è il numero 12 che concerne le funzioni direttive giudicanti di legittimità di semplice presidente della sezione della Corte di cassazione

dei commi che ho citato, peraltro ‑ pure in maniera sintetica - ci dà indicazione di qual è la scelta operata e ci fa capire per quale motivo vogliamo evitare l'intervento dell'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura a questa scelta e a questo *iter* procedurale molto ristretto. Ribadisco i requisiti fondamentali che devono essere valutati, assieme ai requisiti di carattere generale, che sono quelli concernenti, ancora una volta, la capacità scientifica e l'analisi delle norme.

Casson. La questione della individuazione dei requisiti che devono essere applicati dalla Commissione... La senatrice Boccia risulta adesso l'ultima iscritta a parlare. Lo dico perché i colleghi ne tengano conto. La prego, senatrice, *(RC-SE)*. La questione dei requisiti che devono essere adottati dalla commissione per assegnare il conferimento delle funzioni, soprattutto di quelle elevate, è stata una di quelle su cui più ci siamo soffermati nell'esame della Commissione giustizia, data la rilevanza di definire con precisione i criteri di dare quindi una indicazione concreta e rigorosa alla commissione, che riducesse i margini di arbitrarietà della valutazione, senza peraltro ovviamente inficiare l'autonomia e la piena responsabilità del giudizio di quella commissione. Si tratta, però, anche di definire un *iter* procedurale

però riportata ai criteri di fondo sull'individuazione di quei requisiti che la Commissione giustizia ha ritenuto dovessero essere adottati. Questo proprio per consentire che ci fosse una valutazione di merito legata alla specificità e alla diversità delle funzioni, ma che in qualche modo però fossero tutte ricondotte a dei requisiti fondamentali, due dei quali sono quelli che abbiamo individuato:

combina ed equilibra in modo più soddisfacente le due esigenze: fornire i riferimenti chiari e rigorosi ai lavori della commissione per l'*iter* procedurale legato alle differenze e funzioni, senza peraltro

sia dell'assegnazione dei posti ai diversi Gruppi o - come io ho chiesto - almeno alla maggioranza e all'opposizione, sia in relazione al controllo delle schede.

sull'ordine dei lavori non era giustificato se non dal fatto, evidentemente, di richiamare qualche collega al voto. A tal fine, sarebbe bastato chiedere alla senatrice Maria Luisa Boccia, che stava intervenendo prima

ho voluto invitare la Presidenza a far sì che non presti il fianco a questi tentativi maldestri per far

sul fatto che non ci siano doppi voti nel momento della votazione elettronica e non ci sia un abuso di schede - come si suol dire - disattese,

un'abitudine, una dimenticanza e poi magari una prassi quella di alzare la mano e parlare sull'ordine dei lavori una volta indetta la votazione dalla Presidenza, altrimenti tutti lo potremmo fare in qualsiasi momento.

non riesco comprendere le ragioni in virtù delle quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, di un concorso per titoli ed esami orali, tra l'altro svolto dalla stessa commissione ipotizzata per il conferimento delle funzioni di legittimità a regime ordinario. Non riesco a capire quali spese ulteriore possa comportare. Sotto questoprofilo mi piacerebbe anche conoscere la valutazione concreta espressa dal Presidente della Commissione bilancio. Sitrattava di introdurre una valutazione concorsuale per la quota del 10 per cento riservata ai magistrati più giovani, proprio per evitare che costoro arrivassero in Cassazione solo attraverso una valutazione semplice, identica a quella svolta per i magistrati con almeno la quarta valutazione di professionalità, un concorso puramente eventuale, aperto solo a coloro che avevano intenzione di arrivare prima in Cassazione, un concorso che avrebbe comunque consentito un approfondimento più concreto, non esclusivamente basato sulla valutazione dei titoli esattamente come avviene per ragioni di avanzamento per anzianità. Quindi, la possibilità di verificare che quei giovani avessero le capacità e le qualità necessarie, non attraverso esami scritti e orali (quindi una ripetizione), ma attraverso almeno un confronto, un esame orale, che poi alla fine spesso si verifica anche nei concorsi per titoli perché il Consiglio superiore della magistratura ha frequentemente l'abitudine di svolgere audizioni di coloro che sono interessati a ricoprire in un ufficio direttivo le funzioni di legittimità proprio per poter conoscere direttamente, attraverso il confronto diretto, i vari aspiranti. Chiedo al

un magistrato possa svolgere le funzioni di sostituto procuratore, di procuratore aggiunto e di procuratore della Repubblica per tutta la sua carriera o che possa fare il giudice di tribunale, il presidente di sezione e il presidente di tribunale?

quanta incrostazione di potere si crei in capo ad un magistrato che per trent'anni esercita le sue funzioni giudiziarie in un piccolo centro.

in un determinato ufficio probabilmente si crea troppi legami con la città in cui vive, ovvero, in qualche modo, assume un potere che va al di là di quello specifico legato

Dottor D'Ambrosio, se lei prima di fare il procuratore della Repubblica a Milano lo avesse fatto a Brescia e dopo cinque anni fosse tornato a Milano, non sarebbe stato diminuito, ma si sarebbe determinata, non per lei evidentemente, ma in genere per il senso delle istituzioni, una piccola cesura

da Presidente del tribunale a procuratore della Repubblica non perché c'è una vocazione successiva, ma solo perché si vuole un incarico direttivo e quello è a disposizione.

**Il Senato non approva.**

dell'opposizione, hanno chiesto di modificare in parti non insignificanti i loro emendamenti e questo la Presidenza

Perchè l'emendamento, nella nuova formulazione, segue al comma 3. Quindi, va messo in votazione seguendo l'ordine di tutti gli emendamenti che sono stati presentati dai rispettivi colleghi. Non cambia assolutamente niente.

Le riformulazioni sono tali per cui non cambiano la sostanza dell'emendamento. Quindi, se non cambia la sostanza dell'emendamento, è del tutto evidente che l'emendamento deve Se è cambiata la sua collocazione, significa che è cambiato sostanzialmente l'emendamento e questo comporta due questioni. Innanzitutto, la riformulazione è inammissibile perché il senatore Brutti non la può presentare;

apre una nuova finestra"). Senatore Castelli, l'emendamento può essere fatto proprio dal Governo in qualsiasi momento, come lei sa benissimo, e può darsi che ciò avvenga.

3. Interverremo poi nel merito dell'emendamento, giudicandone l'ammissibilità (le anticipo che, a mio giudizio, l'emendamento è ammissibile), e valuteremo e verificheremo se il Governo lo farà proprio o meno o, comunque, sentiremo il parere del relatore sulla nuova formulazione. Mi sembra che stiamo procedendo nel modo più tranquillo e sereno possibile e che garantisca tutti: il presentatore dell'emendamento, lei

colloca la disposizione dopo il comma 3, mi sembra assolutamente pacifico che lei non possa fare altro che metterlo in votazione quando si saranno esaurite le proposte emendative al comma 3. Il punto è tutt'altro: fino a quando questo emendamento non sarà firmato Mastella, ed allora conformemente al Regolamento del Senato troverà ingresso all'esame dell'Assemblea, è un emendamento, signor Presidente (lo dico sin d'ora), che dev'essere considerato inammissibile; se così non fosse, è un emendamento che riguarda nuova materia - la diversa collocazione fisica ne è la testimonianza palese - sulla quale io le chiedo che lei apra un termine brevemente congruo

Brutti. L'eventuale ammissibilità sarà giudicata al momento dell'esame dell'emendamento. Abbiamo stabilito finalmente, dopo una lunga discussione, qual è il momento in cui discuteremo di questo emendamento.

non vorrei risultare pedante, ma siccome lei è un Presidente innamorato della prassi, dev'essere ben chiaro che non stiamo istituendo nessuna prassi, ma che l'emendamento viene accantonato.

Senatore Calderoli, è evidente che la dichiarazione del Governo vale a futura memoria, al momento in cui noi, torno a dire, esamineremo il testo decideremo quale sarà la forma.

Signor Presidente, non so quanto valga il tempo che sto per consumare, però molte volte bisogna anche uscire dalle situazioni con la coscienza di aver tentato fino all'ultimo di introdurre momenti di riflessione e ragionevolezza su questioni che hanno la rilevanza che a tutti appare. Ora, le dichiarazioni testé rese dal ministro Mastella sono la confessione della resa senza condizioni della maggioranza al partito dell'Italia dei Valori, che non è ventriloquo, ma è portavoce ufficiale dell'Associazione nazionale magistrati. *(Applausi dai

che abbia un radicale significato di divisione dei mestieri? Approcciamo allora il problema da altro punto di vista. Vediamo se riusciamo

è il sottosegretario Scotti, il quale, nel corso del dibattito in Commissione, a un certo punto, per convincerci della necessità di rinunciare alla rarefazione dei passaggi di funzione possibili (prima si era detto una volta nel corso della carriera, poi due volte nel corso dell'intera carriera), usò un argomento che mi sembrò

differenziandone il trattamento rispetto a tutti gli altri. Difatti, i magistrati di prima nomina non possono in nessun modo scegliere la sede la sede loro più comoda e devono fisiologicamente saltellare da una funzione all'altra per poter conseguire l'avvicinamento alla stessa. Bene, tale emendamento sostanzialmente stabilisce nei primi dieci anni di carriera, fermo l'obbligo per il magistrato di rimanere comunque almeno cinque anni nella funzione (e a nessuno di voi sfuggirà la ragionevolezza di questa previsione, perché cinque anni sono il tempo congruo, il tempo logico perché il magistrato sì insedi nell'ufficio e impari a svolgere il mestiere che gli viene chiesto di svolgere), fermo questo

Questa era l'idea del sottosegretario Scotti, da lui consegnataci nel corso del dibattito in Commissione; questa è l'idea trasformata in una prescrizione puntuale puntuale sulla quale il voto favorevole di Alleanza Nazionale è ovviamente scontato e sul quale chiedo una riflessione ai colleghi della maggioranza.

*(LNP)*. A questo punto nulla osta dal punto di vista regolamentare, ma il significato politico è profondo, perché, diventando un emendamento del Governo, vince il ministro Di Pietro. Quindi, in questa partita, Di Pietro uno, Mastella zero - questo è il dato

poi, all'ultimo momento, arriva il primo Ministro che passa, impone il suo *diktat* e cambia tutto. Ebbene, per i commissari, soprattutto per quelli della maggioranza che si sono dedicati molto a questo lavoro, va tutto bene così? subisce un'altra umiliazione; oggi ne abbiamo subite tante, però questo va bene. Che resti allora agli atti che almeno noi della Lega non ci stiamo: non vogliamo essere umiliati e denunciamo questo modo di agire.

dovrebbe mancare. L'emendamento del senatore Massimo Brutti non so da dove scaturisca, chi l'abbia suggerito, però viene a confortare tutte le tesi, anche della vecchia riforma Castelli, secondo cui un minimo di condizionamento ci deve pur essere. Consentire liberamente un passaggio da una funzione all'altra può far sì che un magistrato requirente si trovi a giudicare, nel caso del penale, lo stesso caso che aveva valutato precedentemente. Prevedere quantomeno che ci sia un distacco da un distretto all'altro, quanto meno il passaggio come prevede l'emendamento Brutti, può essere ragionevole. Verrebbe da dire che

porta a casa un risultato a bassissimo prezzo e poi il Governo sarà salvato un'altra volta.

Capisco che, per l'ora tarda e per l'intendimento della maggioranza, è difficile passare da una «legge Tarzan» ad «emendamenti Tarzan», come quelli che ci accingiamo a votare domani mattina. Il punto politico della vicenda è la grande delusione di questa occasione mancata. Ho sentito con grande preoccupazione che un ministro della Repubblica, il ministro Di Pietro, ha detto che lui sta con i magistrati. Noi, purtroppo, stiamo con il popolo.

proprio perché esso si propone di venire incontro, in un clima costruttivo e assolutamente utile a realizzare un contemperamento di diverse soluzioni, alle indicazioni provenienti dal sottosegretario Scotti nel corso

in un numero minimo le possibilità di cambiamento di funzioni, in quanto spesso l'avvicinarsi alla sede agognata comporta necessariamente un mutamento di funzioni. Si è allora ipotizzata la possibilità che, per i primi dieci anni di esercizio delle funzioni, non vi fosse alcuna forma di limitazione quantitativa della possibilità di passare da una funzione all'altra, proprio per agevolare l'avvicinamento alla sede agognata.

sede ogni tre anni in Italia. Ma i magistrati tengono famiglia; si devono avvicinare a casa e devono far sì che la moglie lavori vicino casa. Gli altri sono, ovviamente, una razza diversa e separata e seguono necessariamente questo *tour*,

tale possibilità, ipotizzando che successivamente fosse possibile soltanto un cambio di funzione. Se un cambio viene ritenuto troppo esiguo, si può arrivare a due cambi (così come un emendamento successivo recita); si consideri però che, alla fine della storia, se si ipotizzano due cambi dopo i primi dieci anni, si arriva ai famosi quattro, che poi non si verificheranno quasi mai nell'arco dell'intera carriera di un magistrato. A me pare che ci troviamo di fronte ad una norma simbolica; è una norma simbolo quella che si vuole lanciare. Non so quali siano diventati i portavoce dell'ANM e del CSM, portavoce istituzionale a sua volta dell'ANM, perché stati fatti e le indicazioni fioriscono e quindi si sta ampliando la platea di questi portavoce. Se ve ne sono - e probabilmente ve ne sono - penso che agiscano con una certa miopia politica. miopia politica perché pensano che quello sia il luogo dominante e l'organismo di maggiore potere, forse perché ricevono anche sollecitazioni, condizionamenti, messaggi. Allora, è evidente che la miopia farà sì che questo salire su un carro di un vincitore solamente fittizio e temporaneo verrà meno nella prossima legislatura, quando la volontà popolare si esprimerà e farà sì che non vi possano essere più condizionamenti di alcun tipo e scioperi scioperi condizionati ad un eventuale mutamento del testo proveniente dalla Commissione all'esame dell'Aula. Lo sciopero, tra l'altro, è assolutamente ridicolo nell'indicazione della data: tutti sanno che dal 18 luglio in poi udienze non se ne faranno nel modo assoluto; c'è una circolare dello stesso Consiglio superiore della magistratura che le fa concludere al 15 luglio, proprio per far sì che vi possa essere un assorbimento dell'arretrato. È uno sciopero, quindi, assolutamente inattuabile inattuabile che vedrebbe comunque a casa i magistrati. Tale opposizione a questo, ma anche ad altri emendamenti che addolciscono, sotto il profilo quantitativo, questa limitazione, a tutta evidenza dà ragione a chi ritiene e continua a sostenere che vi sia un convitato Di Pietro - chiedo scusa,

di valori o addirittura di chissà quali etiche o di chissà quali impossibilità di toccare autonomie e indipendenze. *(Applausi dei senatori

perché in questa maniera non viene messa l'Aula in condizioni di votare su alcunché. Questo è solo l'*incipit* dell'emendamento, non indica la volontà; sarebbe come se io presentassi un emendamento in cui dico di sopprimere le parole «i magistrati ordinari», punto.

disciplina presente nella norma proposta dalla Commissione all'Aula (mi riferisco agli emendamenti 2.138, 2.139 e 2.142), con gli altri emendamenti si tocca esclusivamente il numero delle volte indicato nella previsione proposta dalla Commissione all'Aula, quindi non vi può essere una decadenza e una preclusione di questo genere di emendamenti, così come lei ha elencato, fino al 2.145.

respinta, decadrebbero. Analogamente avviene per la seconda parte, che noi metteremo in votazione evidentemente se la prima parte venisse ad essere approvata. una logica conseguenza, è la prassi che abbiamo costantemente seguito e mi dispiace che il senatore Caruso abbia fatto riferimento ai precedenti della Presidenza del senatore Mancino, che sono esattamente stati seguiti dalla Presidenza del senatore Pera per tutta la scorsa legislatura. È una prassi consolidata. Mi meraviglia che facciamo delle discussioni come quella che poc'anzi abbiamo fatto su prassi consolidate e anche su logiche che dovrebbero guidare la nostra

contesto anch'io l'interpretazione che ella ha dato dichiarando che sono preclusi tutti gli emendamenti fino al 2.145, perché se lei mette in votazione la parte relativa al «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera», lei obiettivamente

non può dichiarare preclusi gli emendamenti che sono stati presentati che prevedono di sostituire la formula quattro volte con due volte o con tre volte, perché sono emendamenti di portata modificativa radicalmente diversa.

Quindi, l'interpretazione che abbiamo dato di questa procedura è assolutamente corretta. Insisto. Ho chiesto i precedenti ai funzionari del Senato e domani, a scanso di equivoci di ogni genere e tipo, forniremo notizie ai colleghi che hanno sollevato la questione.

tre passaggi di funzione nei primi dieci anni ed un passaggio dopo dieci anni, cioè sostanzialmente siamo di nuovo a quattro passaggi con l'unica differenza rispetto al testo varato in Commissione che se un determinato soggetto, perché ultimo in graduatoria, è costretto ad andare, ad esempio, ad Aosta e vive ad Agrigento, può utilizzare nei primi dieci anni i tre trasferimenti di riavvicinamento e poi decidere dopo i dieci anni cosa fare da grande. Allora, al di là dei tabù, mi pare un emendamento estremamente sensato, che va realmente in favore dei magistrati, perché valuta in maniera positiva le difficoltà di riavvicinamento alla sede di provenienza. Credo non vi sia davvero nulla di male se se ne sospendesse la votazione oggi e, pur rendendomi conto che non è un problema politico per cui può cadere il Governo in ragione in ragione delle diatribe tra il ministro Mastella e il ministro Di Pietro, credo vi possa essere un approfondimento della maggioranza e, se proprio lo dovete respingere, lo potrete fare domani.

**Il Senato non approva.**

prospettare all'Assemblea una soluzione, a mio avviso, equilibrata, che ci aiuta a lavorare più tempestivamente. Premetto che, poche ore fa,

credo che si sia nelle condizioni di poter lavorare risparmiando tempo sulla base di una decisione che è stata responsabilmente assunta in Aula dal ministro Mastella. Non ho alcuna difficoltà ad accettare il fatto che l'emendamento da me presentato e, coerentemente alla valutazione complessiva che da esso emergeva, riformulato,

altro che portavoce, e poiché si vuole esprimere simpatia nei confronti dell'uno o dell'altro intervento dei colleghi dell'opposizione, voglio esprimere la mia simpatia per l'intervento del collega Centaro che diceva che «l'emendamento addolcisce». Mentre il collega Caruso immagina ventriloqui che fanno parlare altri a nome loro, il collega Centaro con

in primo luogo, a differenza di quanto lei ha annunciato, in Aula è presente un testo 3 di questo emendamento, che è stato distribuito, non siamo a quel testo

emendamento evidentemente cambia radicalmente, con l'inserimento di una serie di impedimenti, tutta la procedura relativa al mutamento di funzioni, anche con riferimento al testo 1

Per avere uno scontro con l'opposizione? Se questa è la *ratio*, d'accordo, ne prendiamo atto, ma non vi è alcuna motivazione di natura tecnica per fare ciò. La mia proposta è: domani mattina l'emendamento, abbiamo tempo un paio d'ore affinché gli Uffici, su nostre indicazioni, possano presentare i subemendamenti e lo votiamo. Non vedo quale problema ci possa essere su questa strada.

perché l'intervento del senatore Brutti, da questo punto di vista, mi sembrava riproporre un problema che invece era stato risolto. Ne parleremo e decideremo domani mattina, ma domattina parleremo, decideremo e subemenderemo - se ho capito bene - l'emendamento del Governo,

Facciamo questa precisazione in maniera tale che anche sotto il profilo politico - credo sia nell'interesse sia della maggioranza che dell'opposizione - si sappia che a questo punto l'emendamento del quale stiamo discutendo è un emendamento del Governo.

finestra"). Posso dirle subito, collega Morando, che questa Presidenza avrebbe considerato assolutamente ammissibile - e non aveva il benché minimo dubbio - l'emendamento presentato, ancorché corretto all'inizio della seduta, da parte del senatore Brutti. questo in risposta al senatore Castelli dal momento che, anche soltanto nel corso del dibattito che abbiamo fatto sull'ordinamento giudiziario, su tutte le norme che sino adesso abbiamo esaminato, ripetutamente colleghi, sia di maggioranza ma soprattutto di opposizione, hanno apportato agli emendamenti da loro stessi presentati delle modifiche significative che sono state consentite dalla Presidenza.

ha fatto qui una dichiarazione estremamente precisa, senatore Centaro, dicendo che faceva proprio integralmente

Alle ore 9 si terrà la Conferenza dei Capigruppo e, successivamente, potremo valutare, all'inizio della seduta, se iniziare la discussione

si parla di interpretazioni regolamentari ed è anche un fatto culturale, oltre che piacevole. Tuttavia, Presidente, a parte gli arzigogoli che possono servire per avvantaggiare questa o quella tesi, questa o quella parte,

è stato detto che quell'emendamento era stato ritirato e lei stesso ha riconosciuto che tale affermazione era stata impropria e le devo dare atto di questa sua grandissima disponibilità: in effetti, l'emendamento era stato riformulato.

modo l'emendamento, hanno fatto riferimento alla possibilità del Governo di presentarlo e farlo proprio. Il ministro Mastella, che è un esperto di regolamenti parlamentari, ma che secondo me, in quella fase, ha sentito il dovere di risolvere il problema per il buon andamento dei nostri lavori, giustamente, indotto da questo dibattito, si è alzato ed ha dichiarato di far proprio l'emendamento, come per dire «tagliamo la testa al toro e risolviamo il problema!».

e che essa è ammissibile, personalmente ritengo che non potesse fare diversamente, perché, dopo tutte le riformulazioni a cui abbiamo assistito da un anno a questa parte all'ultimo secondo

Vi è stata poi una difficoltà di collocazione e a questo riguardo è nata la stessa discussione: se viene ricollocato in un altro punto del fascicolo, allora si tratta di un a mio avviso correttamente, precisando che siccome la riformulazione, a parte i contenuti, spostava la collocazione dopo il terzo comma,

anche perché, signor Presidente, presentare un emendamento uguale ad un altro già riformulato è sempre possibile, ma in ogni caso l'emendamento del Governo, uguale a quello presentato dal collega Brutti, non lo sostituisce ma tutt'al più lo affianca. non può sostenere un emendamento e farlo proprio, talché di per sé il presentatore di quell'emendamento è costretto a vedersi ritirato il proprio. Il Governo può benissimo far proprio un emendamento, nel senso che ne presenta uno uguale, ma non sta scritto da nessuna parte che quello presentato dal Governo sia sostitutivo di un emendamento riformulato.

una opportuna concessione all'opposizione. Ripeto: un'opportuna concessione all'opposizione. Infatti, se si tratta di una riformulazione i subemendamenti propriamente non sarebbero consentiti.

ma opportunamente ha consentito all'opposizione di presentare subemendamenti. Penso che in modo ragionevole diversamente non potesse essere fatto dalla Presidenza. Ripeto, dai banchi della maggioranza ovviamente avrei chiesto di non concedere il tempo per la presentazione dei subemendamenti. Onestamente però riconosco che il comportamento della Presidenza è stato opportuno

approvo l'operato della Presidenza e la farei finita qui.

Penso che l'emendamento da me aggiustato oggi pomeriggio fosse a pieno diritto una riformulazione, così come lo era l'emendamento presentato dal collega Nitto Palma che spostava l'intero asse della norma in un'altra direzione. Quindi, si trattava di una riformulazione. Tuttavia, poiché a me interessa la sostanza ed oggi sono stato qui a condurre, collega Caruso, una battaglia politica che spero domani di vincere, domani di vincere, il punto chiave è che si vada a votare quell'emendamento, secondo quel testo, valutando tutte le critiche e tutti i subemendamenti possibili, in un tempo possibilmente non troppo lungo. È l'emendamento del Governo? È l'emendamento del Governo. C'è bisogno di un atto formale di ritiro? Si compia un atto formale di ritiro. Il problema è che poi noi dovremo votare. Se per l'opposizione è importante, tanto meglio, perché tutto ciò che contribuisce a rendere più disteso il rapporto fra noi e l'opposizione è utile al nostro lavoro. Quindi, se per l'opposizione ha significato il fatto che l'emendamento in esame sia l'emendamento del Governo, benissimo, che quello sia l'emendamento in esame. A me interessa che esso corrisponda puntualmente, parola per parola, comprese le virgole, come puntualmente corrisponde parola per parola, comprese le virgole, all'emendamento

senatore Malan.

per l'interpretazione di sette parole nell'introduzione della Costituzione degli Stati Uniti vi fu una guerra di cinque anni. La famosa iota che divise la cristianità antica è un altro esempio. Ricordo invece un esempio assai meno solenne ed assai più recente in Aula, dove la maggioranza, su indicazione del ministro Padoa-Schioppa,

che ci fosse una costante attenzione alla forma perché dalla forma possono venire gravi problemi di sostanza. In questo caso, vorrei sottolineare che bene ha fatto, sia pur tardivamente, il senatore Brutti a ritirare il suo emendamento: il Governo ha manifestato l'intenzione di presentare a sua volta un emendamento. Però, innanzitutto necessario l'atto formale e materiale di presentazione dell'emendamento anche perché quello che ho davanti - credo di non essere in questo meno informato degli altri senatori - è un testo 2, firmato da

la presentazione di un emendamento del Governo non poteva essere fatta così alla leggera. Probabilmente le regole sono cambiate, ma non mi risulta che il Governo potesse presentare

ma l'organizzazione interna del Governo, il quale ha già dimostrato nel passato di avere qualche problemino, perché lo stesso segretario del Consiglio dei ministri dimostrò, all'uscita del Consiglio dei ministri, di non sapere di cosa... PRESIDENTE. Non sta mantenendo la promessa, senatore Malan.

ha parlato di concessione fatta all'opposizione. Le parole sono importanti. Se è un diritto - e lo è - presentare subemendamenti ad un emendamento presentato per di più dal Governo durante la discussione, è un diritto e non è una concessione. Il fatto di lasciare esercitare un diritto è cosa lodevole, come lo sarebbe una concessione, ma è un diritto, e non una concessione. E credo che dobbiamo essere attenti anche a questi aspetti.

Penso che l'avvocato Boccia abbia fatto perdere la causa al cliente perché, al di là della lunghezza della sua arringa, che spesso poi infastidisce anche i giudici,

Questa vicenda poteva essere risolta prima, brillantemente, senza dare adito a tante discussioni, solo che non ci si fosse incaponiti in una scelta, decisa o suggerita, assolutamente sbagliata sotto il profilo procedurale. Dovremo però verificare anche la validità formale di questo emendamento sotto il profilo del presupposto che esso possa essere assentito o licenziato dal Consiglio dei ministri. Sotto questo profilo, sarà mia cura verificare se tale procedura è necessaria o meno.

e non, e lo faccio perché lo giudico un collega di valore; il fatto che le sue battaglie possano corrispondere a delle mie sconfitte non è cosa che mi agita tanto. Mi rammarica però il fatto che egli vinca questa battaglia, quella che probabilmente egli effettivamente vincerà domani, perché sarà una battaglia contro i cittadini, contro il Parlamento. Vince solo lui, per il resto perdiamo tutti insieme. Le ho però chiesto la parola, Presidente, per dirle che che posso accettare, in una giornata densa di lavoro, anche quelli che giudico e ribadisco essere suoi gravi errori nella conduzione dell'Aula, con riferimento alla cosiddetta pratica del canguro, ma non posso accettare concessioni dal senatore Boccia e dalla maggioranza tutta. E siccome il senatore Boccia di concessioni ha parlato con riferimento ai subemendamenti che io avevo chiesto fossero consentiti, per quanto mi riguarda - e per quanto ovviamente riguarda solo me - vi rinuncio.

di far proprio l'emendamento. Se invece, come credo, si tratta della presentazione da parte del ministro Mastella di un testo identico, che come tale è stato presentato *ex* *novo* non facendo proprio l'emendamento del collega Brutti, chiedo alla Presidenza di valutare l'ammissibilità del testo Mastella. Infatti, in quanto emendamento nuovo, credo vada un po' disillusa la prassi che abbiamo introdotto al Senato e che invece appartiene alla Camera, per cui Governo e Commissione possono presentare gli emendamenti Così non è e non è previsto. Qualunque emendamento può essere presentato anche da parte di un senatore, se la Presidenza lo ammette. In attesa di questa valutazione, faccio mio

integrato, di cui era prima firmatario il senatore Brutti. Ho già detto e ribadisco che non avevo il benché minimo dubbio sul considerare quel testo ammissibile e discutibile da parte dell'Aula. Su tale testo, non per una concessione a chicchessia, ritenevo corretto, data la rilevanza della materia e il punto fondamentale che con esso discutiamo,

Quindi, secondo questa Presidenza, era fuori discussione - lo ripeto ancora una volta - l'ammissibilità dell'emendamento di cui era primo firmatario il senatore Brutti con le ultime correzioni apportate nel corso della seduta di oggi; così come sono state ritenute ammissibili correzioni significative di emendamenti presentati da colleghi di diversi Gruppi parlamentari

Sino a quel momento, lo dico anche al senatore Calderoli, la Presidenza aveva sul tavolo esclusivamente l'emendamento del senatore Brutti. del senatore Brutti. dalla prima all'ultima parola a quello del senatore Brutti, di cui è firmatario il ministro Mastella, a nome dell'intero Governo. Il Governo ha formulato ed ha presentato un emendamento identico nella forma e nella sostanza a quello presentato dal senatore

In base alla presentazione dell'emendamento da parte del Governo, al senatore Malan vorrei dire che sono poi problemi del Governo... Non le impedisco assolutamente nulla; può far suo l'emendamento. Ci sarà anche un emendamento Calderoli identico a quello del Governo, però le assicuro che il Governo ha presentato e formulato l'emendamento. Materialmente l'emendamento c'è, senatore Centaro, e su questa base do facoltà ai colleghi di presentare i subemendamenti entro le ore 9,30 di domani mattina, in modo tale da consentire alla ripresa dell'Aula, se l'Assemblea e

se questa autorizzazione l'ha data lei, ne discuteremo domani ovviamente, ma che sia chiaro: il Regolamento non consente automaticamente che il Governo possa presentare emendamenti in corso d'opera. PRESIDENTE. Il Governo, come lei ben sa, presenta emendamenti quando vuole.

in riferimento all'intervento di questa mattina del senatore Castelli, che è stato da me interrotto certamente in modo intemperante. Per questo, porgo le mie scuse all'Aula. La mia intemperanza era dovuta però a un senso di ingiustizia che incombeva sul Senato, a una mistificazione della realtà. Ho interrotto il senatore Castelli dicendo che non si produce democrazia con i pianisti. Il senatore Castelli ha fatto riferimento ancora una volta al consenso dato da un senatore a vita all'articolo 1 della riforma dell'ordinamento giudiziario che stiamo affrontando. L'esito di quella votazione Ben cinque senatori della minoranza, pur votanti e non avendo il dono dell'ubiquità, non erano in Aula. Grazie ad abili pianisti risultavano però presenti, inficiando quindi il risultato. Era questa l'intollerante ingiustizia che ha portato a uno strumentale percorso politico a cui abbiamo assistito tutti. Il senatore Castelli non ha perso occasione per alimentare offese personali. Oggi in Aula molti colleghi della maggioranza sono stati definiti ventriloqui, servi, schiavi schiavi dei magistrati, lobbisti. Nei miei confronti il senatore Castelli non ha certamente usato parole dolci. Non certo a lui devo rispondere, ma agli elettori che hanno nei miei confronti espresso il loro consenso. È vero che in quest'Aula sono intervenuto pochissime volte, soprattutto per disciplina di coalizione, visto anche l'ostruzionismo che voi della minoranza applicate a pie' sospinto. Ma le assicuro che nelle Commissioni a cui partecipo non mi risparmio.

D'altronde, nel suo intervento in Commissione antimafia, la risultanza di un odio viscerale del senatore Castelli nei confronti del Sud era evidente. Castelli, di cultura lombrosiana, non perde occasione per manifestare queste idee. Ma dall'ex ministro Castelli, secessionista di vecchia guardia, dall'ex Ministro della giustizia, eletto nel Parlamento italiano, che insieme ai suoi leghisti ha calpestato il Tricolore e che qui, davanti Palazzo Madama, ha gridato «chi non salta italiano è», non intendo prendere nessuna lezione, né di cultura, né di politica, né di vita.